Signora Presidente, onorevoli colleghi, vice ministro Vegas, come quella dello scorso anno, anche la finanziaria in esame può essere definita snella. In materia di conti pubblici l'Esecutivo continua ‑ aggiungo opportunamente ‑ sulla strada della prudenza, quella tracciata sin dall'inizio della crisi internazionale, perché, nel perdurare le difficoltà finanziarie ed economiche, non si è fatto trascinare sul terreno, pur lusinghiero e facile, delle politiche di bilancio espansive. Un eufemismo, quello dell'espansione, che si sarebbe tradotto in faraonici programmi di spesa, in deficit certamente, magari tutt'altro che anticiclici e - aggiungerei - che tutti poi avremmo pesantemente pagato. Il Governo invece ha preferito mantenere un profilo basso, nel rigore riconosciuto positivamente nel dibattito dagli economisti, riproponendo la politica dei piccoli passi, quella delle misure e della tutela del risparmio e del sostegno ai redditi. Misure efficaci e non onerose, in qualche modo non popolari, forse, perché non roboanti, ma che hanno evitato le tensioni e gli scossoni sociali, ancor più di quelli economici che si sono registrati invece in altri Paesi. Il Governo ha scelto di garantire la stabilità dell'intero sistema, in una parola. Certamente la crisi non ci è alle spalle e i fenomeni che ne sono scaturiti contengono una vischiosità che potrebbe mostrare gli effetti più in là; tutti da registrare e da valutare attentamente, ma ad oggi - e non si può dire che di tempo non ne sia passato - il Paese sta reagendo meglio di quanto previsto agli inizi del 2008; e mi sembra un'affermazione non avventata, ma anzi supportata dai dati contenuti nei documenti di istituti e istituzioni economiche. Ad esempio, nelle più recenti previsioni, la Commissione europea stima per il prossimo biennio una crescita del nostro PIL ulteriormente migliorativa di quella fornita in estate. Peraltro, vale la pena ricordare che il nostro ad oggi è un PIL migliore persino di quello della Gran Bretagna e fornisce elementi incoraggianti anche, come la sostanziale tenuta della disoccupazione e l'incremento dei consumi privati. Pur con tutte le difficoltà, l'indice della nostra produzione industriale ha recentemente fatto registrare un significativo balzo in avanti, così come quello della fiducia dei consumatori calcolato dall'ISAE, che appare salito al punto più alto dal dicembre del 2006, prima Mi guardo bene certo dall'alternare rispetto a questi dati che tutto va per il meglio; dico solo che esiste una certa robustezza del settore privato, di quello creditizio e di altri settori che tengono meglio di quello tipicamente industriale. Insomma, una complessiva solidità del sistema, che forse è alla base del giudizio favorevole recentemente espresso da Moody's sul debito pubblico dell'Italia, nonostante questo sia purtroppo in crescita nel prossimo biennio.

significa che esso ha saputo ben operare in una situazione di emergenza? Che è superato l'*unfit* che «The Economist» appioppò al Presidente del Consiglio? Sono convinta che sia ma tutto ciò non significa che da parte del Governo e di questa maggioranza manchi la consapevolezza che oggi va preparata la ripresa e che occorre dare la spinta con nuove misure per il rilancio economico e sociale. nel corso dell'esame in Commissione sono stati molti gli spunti che, al di là delle modifiche al testo originario, portano a questa conclusione: dalla revisione quantitativa e qualitativa della spesa alla possibilità di ridurre il carico fiscale sulle imprese con una manovra seppur limitata sull'IRAP. Tale manovra a mio avviso potrebbe articolarsi in un meccanismo che ne eviti l'applicazione alle imprese che sono in perdita (ricordo che oggi pagano l'IRAP sia le imprese che producono utili sia quelle che sono in perdita) oppure individuando un meccanismo di deducibilità, peraltro già oggetto di diversi disegni di legge anche da me presentati.

con la quale vengono destinati 10 milioni di euro agli interventi in favore dei consorzi Confidi delle Province che - non a caso - presentano il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione guadagni. Se è vero - come credo che sia - che la partita che si aprirà nei prossimi mesi nell'ambito della ricaduta della crisi economica sull'economia reale riguarda la tutela dei lavoratori e la patrimonializzazione delle imprese, in entrambi i casi il Governo sta agendo bene, rafforzando il sistema della cassa integrazione e offrendo alle imprese solidi strumenti per consolidarne la tenuta sul sistema finanziario, nella preoccupante prospettiva di Basilea 2. 2. Piuttosto che il vecchio armamentario dei fondi agevolati, è arrivato il momento di pensare a strumenti più moderni ed efficaci per le imprese, che dovranno affrontare la ripresa, sostenuti da fondi di garanzia che permettano loro di accedere a quel credito che si è fatto più difficile per i vincoli stringenti del sistema bancario, che spesso non condividiamo. Penso però anche al nuovo soggetto societario Difesa servizi Spa, ente *in* *house* del Ministero della difesa, che può costituire una modalità operativa nuova per la pubblica amministrazione, non solo dal lato dei costi, ma anche da quello dei ricavi, in termini di valorizzazione economica delle proprie risorse. Sono sicura che il Senato lavorerà in questo senso migliorando ulteriormente lo strumento, perché diventi una possibile forma di autofinanziamento per l'amministrazione, che nello specifico non significa solo operatività simile a quella di CONSIP, ma valorizzazione dei servizi forniti. vale per la proroga del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti, detenute storicamente in banche popolari: si tratta di una disposizione resa necessaria dal protrarsi della situazione di difficoltà dei mercati e dall'andamento negativo dei corsi azionari, che evita di effettuare consistenti svalutazioni ai detentori delle partecipazioni stesse. La consapevolezza che non possiamo contraddire le misure efficaci e non onerose intraprese fino ad oggi ci porta a dire che è necessario ora liberarci di dirigismi di varia natura e di appesantimenti fiscali iniqui e controproducenti, ma anche di ridurre la spesa per consentire il sempre presente obiettivo della riduzione della pressione fiscale. Ha ragione il senatore Massimo Garavaglia quando ricorda che forse è la prima volta che in questa Camera si è lavorato sulle possibilità e sulle modalità di taglio alla spesa, piuttosto che sull'aumento delle tasse. In fondo, restiamo fedeli all'idea che sia necessario aumentare il prodotto nazionale senza creare un nuovo debito pubblico, e al Governo Berlusconi va il merito di essere coerente con gli impegni assunti davanti agli elettori italiani efficace più di altri Governi europei in questa difficile situazione economica. Gli italiani lo sanno, e con il loro consenso determinano il nostro convincimento ad andare avanti e a proseguire su questa strada. *(Applausi

per formulare un giudizio intellettualmente corretto ed onesto sulle proposte della legge finanziaria, penso che dobbiamo riflettere sul contesto assai difficile, di cui occorre essere consapevoli. Pochi dati sono sufficienti. Con riguardo al PIL, gli ultimi dati per il consuntivo 2009 variano tra il meno 4,8 della relazione previsionale ed il meno 4,7 delle ultime previsioni UE. Dobbiamo essere consapevoli di cosa significa questa perdita drammatica di ricchezza del Paese: vuol dire che se l'Italia crescesse al ritmo in cui è cresciuta negli ultimi 10 anni ci vorrebbero 15 anni per tornare al livello di ricchezza del 2007. Relativamente all'occupazione, sono circa 650.000 i posti di lavoro persi, non solo nel lavoro dipendente, ma anche nell'area del lavoro autonomo e, soprattutto, precario. Più di 1 milione di cittadini in questi momenti sono interessati o dalla perdita del lavoro o dalla sua incertezza (cassa integrazione e mobilità), e tutti gli indicatori segnalano che la situazione è destinata ad aggravarsi nel 2010, pur scontando un miglioramento della congiuntura. Il problema è che i magazzini sono pieni; si stanno esaurendo gli ammortizzatori sociali, ci sono chiusure di aziende travolte dal troppo lungo e pesante ciclo negativo. L'*export* è calato del 23,6 per cento, mentre la produttività del manifatturiero italiano è calata in un anno di oltre tre punti. La pressione fiscale a fine 2009 è stimata al 43 per cento: è la più alta pressione fiscale dal dopoguerra, tranne l'anno di entrata nell'euro, con l'aggravante che è aumentata la tassazione sul lavoro dipendente e la tassazione sul contribuente leale. La spesa pubblica ha raggiunto il *record* del 52,4 per cento del PIL, il più elevato negli ultimi cinquant'anni, con una crescita di tre punti in un solo anno. E cresce la spesa dello Stato centrale, più di quella decentrata; cresce la spesa per il funzionamento della macchina burocratica, più che quella per gli investimenti. Il ministro Brunetta avrà usato slogan efficaci, ma il fatto è che quest'anno la macchina dello Stato ha assorbito più risorse dell'anno precedente. Il debito supera il 114 del PIL, con un incremento di nove punti percentuali. Volendo continuare nelle mie citazioni mozartiane del Don Giovanni, potrei dire che «il catalogo è questo», come dice Leporello a Donna Elvira, ma è un catalogo difficile, difficile, pesante. Però nasconderlo o sottovalutarlo è la cosa peggiore. Il Governo ha fatto una scommessa che si è rilevata sbagliata. Ha pensato che la crisi sarebbe stata meno pesante e meno lunga e che sarebbe stato sufficiente aspettare, adottando nel breve un po' di cosmesi politico-finanziaria. Non ha valutato che questo pesante quadro congiunturale si sovrappone a limiti strutturali di competitività del sistema Paese e che la somma di queste due componenti dà per risultato non una parentesi da aprire e chiudere per tornare come prima, ma richiederebbe una forte azione per rimediare ai ritardi con riforme coraggiose. Il largo consenso parlamentare del Paese, di cui si vanta un giorno sì e l'altro pure il Presidente del Consiglio, avrebbe dovuto a nostro avviso produrre un'agenda riformista su cui sfidare l'opposizione, e noi avremmo accettato volentieri questa sfida virtuosa. Una politica con l'orgoglio di vincere davvero una sfida storica per rimediare ai ritardi del Paese; una sfida su cui costruire alleanze sociali. Dov'è questa agenda riformista ? Non certo in questa legge finanziaria e neppure nei farraginosi provvedimenti che si sono stratificati nel corso dell'ultimo anno. Esiste un lancio giornalistico di riforme, come se queste fossero un bene di largo consumo, ma non ci sono i fatti. Basta qualche esempio. Quando, se non ora, il tempo di una riforma strutturale degli ammortizzatori sociali? Ora, che una drammatica pressione sociale sulla disponibilità di lavoro può portare tutte le forze responsabili a condividere un'impostazione più larga, più equa, più efficiente, nell'interesse del Paese. Le nostre proposte le abbiamo messe in campo; il Governo non ha avuto il coraggio di seguire questa strada. È un capitolo difficile, certo, ma quando i tempi sono difficili i compiti della politica sono più difficili. Quando, se non ora, sarebbe necessario impostare una solida *spending review* del bilancio per agire sull'inefficienza della spesa, non con annunci qualunquistici e inconcludenti, ma con un rigoroso esame della produttività della spesa pubblica? Basta andare ai tanti documenti ed alle tante proposte della Commissione sulla spesa pubblica che il Governo ha irresponsabilmente soppresso. Quando, se non ora, bisognerebbe affrontare quelle riforme, a costo zero dal punto di vista finanziario, che riguardano le aperture dei mercati e il disboscamento degli oneri burocratici per le imprese? Che dire del fisco? è la visione fiscale della maggioranza, oltre la promessa di ridurre la pressione fiscale, cui ha naturalmente corrisposto nel mondo reale un suo aumento? Ora sembra che si interverrà in modo più o meno simbolico sull'IRAP. noi siamo pronti, abbiamo presentato i nostri emendamenti e le nostre proposte. Ricordo che poi l'unica riduzione strutturale e permanente dell'IRAP è stata fatta dal Governo Prodi,

al di fuori di un disegno chiaro di riforma e in un orizzonte di incertezza per le famiglie e le imprese? Sappiamo quali sono i difetti del fisco su cui lavorare: un fisco troppo concentrato sul lavoro dipendente e imprenditoriale e molto poco sulle rendite; un fisco troppo complicato e presuntivo, con la deformazione degli studi di settore; un fisco troppo centralizzato, con una scarsissima relazione tra prelievo e servizi restituiti al territorio. Si è vista una correzione di queste debolezze? Dove, quando? L'unica correzione fatta riguarda qualche strizzata d'occhio per tollerare il ritorno a pratiche elusive ed evasive. Abolirete l'IRAP, sia pure in un tempo incerto e lontano? Bene, Bene, ma com'è possibile fare sul serio una riforma in favore del federalismo fiscale se si abolisce una buona parte dell'ICI, imposta che dava autonomia fiscale ai Comuni, e l'IRAP, che finanzia buona parte dei bilanci regionali? Dire che si abolirà senza chiarire dove si reperiranno le risorse necessarie - e parliamo di 40 miliardi di euro, di cui 27 per la parte privata - e senza dire come si rafforza e non si indebolisce l'autonomia regionale è solo un espediente mediatico di un Governo a corto di idee e di argomenti. Segnalo che intanto si sono già accumulati i primi ritardi per il federalismo.

Il Paese non ha bisogno di espedienti, signori del Governo e della maggioranza: ha bisogno di riforme coraggiose. Sono quelle che continuano a mancare; sono quelle che noi ci ostiniamo a riproporre in ogni occasione.

permettetemi anzitutto di notare un fatto politico importante che è avvenuto in questi giorni, sia in sede di Commissione, sia in quest'Aula, nel corso della discussione generale Colgo l'occasione per ringraziare tutti i membri della Commissione finanze e tesoro che ho l'onore di presiedere, hanno partecipato alla discussione per trasmettere il nostro rapporto alla Commissione bilancio, sia tutti i colleghi della Commissione bilancio, di maggioranza e opposizione, perché il fatto politico da non sottovalutare è che - e non succede troppo spesso purtroppo - si è discusso nel merito, con valutazioni diverse, con contenuti concreti,

questo metodo rappresenti un valore da sostenere e difendere in qualunque momento, anche in termini di rapporto tra Governo e Parlamento

una manovra di bilancio, una politica economica, occorre quantomeno capire e possibilmente concordare su quale sia il riferimento concreto e reale rispetto al quale la manovra intende produrre i propri effetti.

punto di credibilità) che parla di un andamento del ciclo economico internazionale chiamato a "V": cioè, dopo la pesante crisi produttiva in termini di PIL del 2009 dovremmo vedere una ripresa piuttosto consistente dell'economia mondiale nel 2010. Tuttavia, negli ultimi giorni già qualcuno negli stessi Stati Uniti d'America e sui mercati finanziari ha posto un quesito che non va sottovalutato.

nuova e pericolosa. si tratta di *recovery* o di *bubble.* Si tratta di un elemento da tenere sotto controllo per valutare cosa possiamo fare. Ma, anche ammesso che ci sia una ripresa internazionale e che non sia la ricostruzione di una bolla speculativa (i dati sui derivati cominciano già a preoccupare); ammesso che questa ipotesi ottimistica si realizzi nel 2010, qual è la conseguenza sull'economia italiana che, come sappiamo, per due terzi dipende dall'esterno, qualunque sia il Governo nazionale, qualunque manovra esso possa impostare? Due terzi dell'andamento dell'economia italiana dipendono da questo quadro esterno dell'economia mondiale e di quella europea. considerazione questo effetto esterno sull'andamento inerziale tendenziale dell'economia italiana, certamente vediamo che i segni di ripresa appaiono anche per l'economia italiana.

le condizioni economiche, sociali e occupazionali che avevamo prima di cadere nel pozzo della crisi nel 2007. Da questo punto di vista, possiamo anche girare in mille modi i numeretti dell'economia o dell'econometria, ma sappiamo che questa sarà una ripresa lenta, difficile e che ricostruirà i dati del 2007 non prima del 2013-2014. Sappiamo che le condizioni finanziarie della finanza pubblica italiana vanno assolutamente salvaguardate nei loro equilibri: follia e demagogia sarebbe mollare la guardia sul fronte degli equilibri finanziari. Sappiamo, però, che quegli equilibri rimarrebbero relativamente fragili, perché il rientro dal deficit sarebbe relativamente lento ma, soprattutto, perché il rientro dal debito, quel rapporto tra debito e PIL che nel 2007 era era pari al 105 per cento del PIL (quindi già abbondantemente sopra il totale del reddito nazionale), potrà tornare a quel livello, negli andamenti tendenziali e inerziali, intorno al 2020. Nel frattempo, tre gravi rischi incombono sulla nostra economia e sulle nostre condizioni socio-economiche. Il primo, che ho già citato,

potrebbe non proseguire dopo il 2010. Il secondo rischio è che, laddove la ripresa proseguisse in modo strutturale, al primo apparire di eventuali segnali inflazionistici potrebbe esserci una ripresa in aumento dei tassi di interesse. interesse. Per un Paese con il nostro debito ciò significa il rischio di dover pagare molto di più in termini di oneri finanziari sul debito pubblico. Sappiamo già oggi, a bocce ferme e con le informazioni noi dovremmo pagare nei prossimi anni un importo per interessi, che attualmente si aggira intorno a 75 miliardi di euro, che andrà progressivamente a crescere fino a sfiorare i 100 miliardi di euro nel 2013. Questi sono i dati che, con grande trasparenza e correttezza intellettuale, il Governo ha inserito nel DPEF

è che se prosegue l'illusione americana di aggiustare le proprie questioni interne svalutando ulteriormente il dollaro, al quale è agganciato lo yuan cinese (quindi con una doppia svalutazione dollaro-renminbi), ciò comporterebbe una ulteriore ipervalutazione dell'euro fino a 1,60 o 1,70 (e siamo già a 1,50 rispetto al dollaro). Tutto questo creerebbe condizioni di nuova emergenza. emergenza. Questi andamenti tendenziali inerziali ci possono soddisfare e mettere al riparo? La mia risposta è no. Qui va chiarito un punto. Che cos'è, allora, la politica economica, quella vera, concreta, che abbiamo discusso nelle Aule delle Commissioni e in questa?

che garantisce l'equilibrio finanziario della finanza pubblica. Non un euro in più di deficit. Seconda domanda conseguente: garantendo questo,

suo passato e con i dati presenti, purtroppo. Ma se allora la politica economica ha la sua centralità proprio garantendo l'equilibrio finanziario, che cosa significa la politica economica vera? Significa andare responsabilmente a valutare se i livelli di spesa e i livelli di entrate, a parità di deficit, possono o debbono essere modificati, responsabilmente, davanti a quest'Aula e davanti ai cittadini che pagano le tasse. Quegli 800 e passa miliardi di spesa pubblica che ogni anno prevediamo sono tutti efficaci ai fini di equità sociale e di crescita economica? Tutti quegli 800 miliardi producono effetti di maggiore giustizia sociale e di migliori condizioni di produzione e di occupazione? Il dibattito non è su come ridurre le entrate e la pressione fiscale. Tema principe del dibattito è come contenere e ridurre quel Moloch della spesa pubblica. Questa è la risposta, che in qualche misura abbiamo tentato di dare anche con un contributo in positivo un emendamento presentato in Commissione, che ha ricevuto la bocciatura tecnica in quella sede e che è stato ripresentato in quest'Aula, con un quadro di riferimento complessivo: meno spesa corrente, meno tasse su imprese e famiglie, più investimenti. Non è una formula magica; non è una valutazione tecnica; è una precisa scelta, nobile - aggiungo - della politica. E accanto ad un'operazione complessiva che eserciti questa scelta, occorre valutare la politica economica così definita sulla sua capacità di produrre effetti migliorativi su quegli andamenti tendenziali inerziali. Evidentemente, infatti, se una politica economica modifica dello 0,1 per cento il PIL o dello 0,08 per cento l'andamento dell'occupazione, per quanto ragionevole, per quanto rispettabile, non è una politica economica; è un'accettazione degli andamenti tendenziali inerziali. È evidente che quest'opera, che deve far assumere un atteggiamento fermo alla maggioranza e al Governo - ma io credo anche

di quegli 800 miliardi di cui, sulla base delle mie valutazioni e informazioni, almeno il 10 (80 miliardi) non ha nulla a che vedere con la giustizia sociale e con la crescita economica e occupazionale del Paese, ma ha a che vedere con altre cose, con altre faccende. È ovvio che a quella entità di spesa sono interessati, da una parte, varie decine di migliaia di cittadini, di organizzazioni, di consorterie, ma dall'altra anche 57 milioni di italiani. Questo è il peso della scelta politica. È ovvio che non si possa pretendere di fare tutto e subito, ma certamente quell'emendamento complessivo non può che rappresentare la linea guida, la strategia di medio termine di una maggioranza e di un di Governo che di quel triangolo, di quel tridente - meno spesa, meno tasse, più investimenti (e quindi più crescita, più occupazione, più equità sociale) ha fatto, e non da ora, il suo codice genetico politico, sia del Popolo della Libertà sia degli amici della Lega. Lega. Se queste linee guida strategiche sono condivise, occorre capire cosa è possibile ed

che accanto al quadro complessivo abbiamo presentato una serie di emendamenti "monografici" per le imprese, per la famiglia, per gli investimenti infrastrutturali, per le forze di polizia e di sicurezza, per la ricerca scientifica e l'università. È evidente che la quantità di ciò che è possibile fare è tutta da discutere ed è legata in un rapporto «uno a uno» al taglio delle spese. Quindi, se quella è la quantità complessiva che può essere stabilita in quest'Aula pro quota, quello è il pro quota che può essere trasferito nel pro quota della riduzione fiscale a famiglie e imprese e del rilancio e sostegno alla crescita e all'occupazione. Su questo c'è la più totale disponibilità, perché è ragionevole, saggio e di buon senso.

le deduzioni e il coefficiente familiare per le famiglie e così via. Non mi dilungo oltre.

da un possibile equivoco: le entrate dello scudo fiscale, nonché l'andamento dell'autotassazione di novembre sono elementi importanti da valutare nel momento in cui ci saranno, ma non hanno nulla a che vedere con il ragionamento che ho tentato di delineare. Infatti, è ragionevole pensare che se ci saranno entrate fiscali dallo scudo,

con una definizione nota e matematica, che varrebbe la pena applicare qui per la politica, quella che ho ritenuto essere seria, con un confronto aperto e con una disponibilità posizioni di buon senso. Occorre fare questa scelta strategica, occorre definire le quantità, l'entità e la qualità del tridente: parte un percorso delineato, sappiamo dove andiamo a finire, facciamo il primo passo. Occorre qui stabilire il massimo comune divisore, perché nei passi successivi si trovi il minimo comune multiplo. La maggioranza è pronta a sostenere la linea del rigore del Governo, e a contribuire perché essa sia il passaggio verso

assorbe più della metà del PIL, mentre non siamo sicuri - nessuno di noi - assolva al compito di una migliore giustizia sociale e di una maggiore prospettiva di crescita del reddito e dell'occupazione, per noi e per i nostri figli. *(Applausi dal

ampio che c'è stato da ieri fino ad ora meriti qualche riflessione, anche se breve, considerata l'economia del tempo.

Vorrei precisare qualche elemento, rimandando molte valutazioni a quelle contenute nella relazione di presentazione del disegno internazionale certifica che l'Italia e l'Europa escono dalla recessione. Mi sembra che questa valutazione sia stata ripetuta sia dalla maggioranza che dell'opposizione. Ed ancora, che non si prevede alcun peggioramento

prendendo in esame il debito e l'andamento dei conti che nel medio termine ci portano ad essere in una situazione di tranquillità. Quindi, secondo queste valutazioni l'Italia continua a godere di una buona, sufficiente, credibilità, sia in campo fiscale che in quello economico, nonostante l'impatto negativo della crisi. Bisogna, quindi, continuare a far convivere - credo - misure di stimolo e azioni di riduzione del debito.

è una condizione di fatto, che si deve assumere l'intero Paese negli articolati livelli di governo, consapevoli, tutti, che alti livelli di debito ritardano in ultima istanza ogni dinamica di crescita e che alti livelli di debito si associano, peraltro, ad andamenti di bassa crescita e per lunghi periodi, come dimostrano i casi dell'Italia e del Giappone. Il Governo in questo anno e mezzo di legislatura non è stato a guardare: mi sembrerebbe un giudizio ingeneroso. Non solo ha messo in sicurezza i saldi di bilancio - e mi pare che questo giudizio sia condiviso da molti ma ha messo al riparo da conseguenze peggiori il nostro sistema creditizio, con interventi di garanzia per i depositi e di rafforzamento patrimoniale per le banche: Presidente, lo scenario mondiale, il fallimento e la nazionalizzazione di importanti istituzioni finanziarie in grandi Paesi occidentali. È stata È stata salvaguardata la coesione sociale - ed anche quest'obiettivo mi pare largamente riconosciuto - con il finanziamento e l'ampliamento delle misure afferenti agli ammortizzatori sociali, perché tanti lavoratori non rimanessero da soli dinanzi alla crisi dell'economia reale. Poi le misure anticrisi, più di una, contenute nei diversi provvedimenti legislativi collegati alla scorsa finanziaria, che qui vorrei ricordare: il Piano casa; il Patto per la salute; l'adeguamento delle pensioni per migliorare l'equilibrio del sistema pensionistico; il varo della riforma della pubblica amministrazione, da cui ci attendiamo un riordino e - perché no - un risparmio; le modifiche del processo civile, e sappiamo quanto pesi in termini di sviluppo la giustizia civile nel nostro Paese; l'avvio del federalismo fiscale; il provvedimento in materia di energia, per contrastare la dipendenza del nostro Paese e mettere mano alla bolletta energetica, che pesa in termini significativi sul sistema produttivo italiano.

sul reddito e sulla produzione di ricchezza dei contesti di riferimento. Da ultimo, vorrei ricordare per il Mezzogiorno lo sblocco dei FAS, di cui spesso abbiamo parlato ed il tentativo di un loro coordinamento per evitare la polverizzazione della spesa e che questa prevalesse sulla finalizzazione verso gli obiettivi del potenziamento della rete infrastrutturale e dell'apparato produttivo. l'avvio del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, richiamato più volte, per un primo modulo di 18 miliardi, operazione inclusa nell'ultima manovra di assestamento, che ha rappresentato un'iniezione di credito per il sistema delle imprese che sicuramente soffrono ed hanno sofferto in questi anni la lentezza e l'arretrato dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche. il sostegno di alcuni settori - come quello dell'auto - che hanno un peso nell'industria italiana ed un impatto occupazionale in molte Regioni del Paese. Per tutto questo - e si tratta solo di alcuni riferimenti - ci sembra davvero ingeneroso valutare o accusare di immobilismo il Governo Berlusconi, il ministro Tremonti e le sue azioni in campo economico.

del centrosinistra, infatti, hanno sottolineato la bontà degli interventi, la fermezza e la prontezza degli interventi del Governo in questa crisi, in particolare nell'ultimo anno e mezzo.

ma purtroppo non ha risposto, alla domanda che avevo cercato di sintetizzare nella mia relazione introduttiva: la politica economica e di bilancio deve rimanere (grosso modo, naturalmente) quella che ha trovato espressione nella legge finanziaria e nella legge di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri, oppure nella politica economica e di bilancio deve intervenire una correzione, nel senso

per realizzare interventi di riequilibrio sociale e di sollecitazione della crescita economica? Questa è l'alternativa che abbiamo di fronte.

Sostanzialmente si tratta di questo: l'economia globale - dice il Governo ed è vero - sia pur in quel contesto di incertezza sulle dimensioni e sulle caratteristiche della crescita di cui si è detto; tuttavia, l'economia globale ha toccato il punto di minimo nel processo di recessione e adesso sta rimbalzando verso l'alto. Questo - dice il Governo - consentirà una ripartenza dei consumi all'interno dell'economia globale; noi - continua il Governo - siamo un Paese produttore di beni e servizi di alta qualità alta qualità e in larga misura esportatore e la ripresa dei consumi alla dimensione globale consentirà finalmente alle nostre imprese, manifatturiere in particolare, di riprendere la produzione a pieno ritmo le esportazioni risaliranno. Per questa via, torneremo su di un sentiero di crescita stabile e duraturo, a condizione conclude sempre il Governo - di non fare scelte di bilancio eccessivamente espansive che allarghino troppo il deficit, in un contesto nel quale resta come una grande minaccia sul sistema Paese (sappiamo quanto questa analisi sia corretta), un volume globale del debito che abbiamo impiegato tanti anni a ridurre da 120 al 105 per cento del prodotto interno lordo e adesso sta risalendo, nel corso di pochissimi anni, nuovamente

(sia pure essendo fondata, ripeto, su analisi che concludono su elementi che, ad uno ad uno, concorrono a formare la realtà che abbiamo di fronte), voglio semplicemente aggiungere due ulteriori considerazioni che dimostrano che purtroppo questa è una rappresentazione autoconsolatoria della realtà. C'è una domanda a cui bisogna rispondere e a cui nessun nessun centro di analisi oggi è in grado di rispondere. Infatti, perché noi, Paese manufatturiero‑esportatore, possiamo tornare a crescere al livello del 2007 e oltre, bisogna che riprendano nell'economia globale a ritmo sostenuto i consumi. Ebbene, nessuno sa in questo momento chi nel mondo nell'economia globale sostituirà le famiglie americane come consumatori globali. tutti sappiamo che l'economia del debito, che ha caratterizzato la fase degli ultimi 10-13 anni, aveva un fulcro ed un elemento di traino nei consumi delle famiglie degli Stati Uniti d'America, la più grande potenza economica globale, per cui si è determinato uno squilibrio in quel Paese, cioè una totale mancanza di risparmio negli Stati Uniti, mentre per altro verso, in Cina, in India, nei Paesi emergenti, si accumulava un gigantesco risparmio, in Cina) e privato, che non incontrandosi con il difetto di risparmio degli Stati Uniti d'America, ha determinato sostanzialmente, dal punto di vista strutturale, il collasso dell'economia globale. la seguente: per rendere realistico il disegno del Governo, chi sostituirà nel mondo i consumatori americani come consumatori globali?

famiglie, se vogliono evitare il fallimento dal punto di vista economico - mi si scusi adesso la forzatura - debbono incrementare significativamente (e lo stanno facendo) il loro tasso di risparmio, in un contesto di redditi particolarmente depressi a causa dell'andamento della crisi e dell'innalzamento della disoccupazione. Altro elemento che cozza nell'economia globale contro l'analisi autoconsolatoria del Governo è che, oltre a non avere consumatori globali, che c'erano e trainavano la nostra capacità di esportazione, c'è un altro grande problema. Prima o dopo - speriamo dopo, ma prima o poi accadrà - i Governi degli Stati Uniti, dei principali Paesi europei, della Cina, dell'India dovranno cominciare a rientrare da quelle politiche monetarie e da quelle politiche di bilancio espansive che sono alla base del fatto che la crisi in quei Paesi ha avuto un effetto tutto sommato non particolarmente devastante e hanno iniziato la ripresa prima di noi. Prima o poi da quella politica fiscale espansiva e da quella politica monetaria espansiva bisognerà che rientrino; speriamo che lo facciano in modo graduale, ma dovranno rientrare. se anche da quel lato avremo una sorta di riduzione della domanda al livello globale, a chi esporteremo i nostri beni, visto che, com'è noto, non ci sono ancora sulla luna compratori che siano in grado di consumare i prodotti italiani, laddove, come si sa sulla base della teoria del commercio internazionale, se c'è qualcuno che esporta bisogna che ci sia qualcun altro che importa? Quindi, non è attraverso l'approccio che il Governo sta considerando come prioritario che noi possiamo sperare di avere una soluzione positiva della grande questione, ovvero come ridurre l'impatto sociale della crisi e come uscirne il più rapidamente e il più solidamente possibile. Quindi, noi abbiamo bisogno di interventi che correggano la politica economica e la politica fiscale nel senso di costruire un *mix* diverso, non nel senso della politica di bilancio espansiva che aumenta solo il deficit: questo non l'ha proposto nessuno e non lo propone nessuno, né nella maggioranza né nell'opposizione. Invece si chiede: è sicuro il Governo che l'attuale *mix* tra politiche di risparmio e politiche di riduzione della pressione fiscale e di aumento della spesa in conto capitale sia quello giusto per fare in modo che l'Italia esca prima dalla crisi e paghi un prezzo sociale minore e, soprattutto, che, una volta uscita dalla crisi, riesca a camminare alla stessa velocità degli altri Paesi nostri competitori?

occorra correggere la legge di bilancio e la legge finanziaria nel senso che ho cercato di indicare all'inizio. I colleghi del mio Gruppo che sono intervenuti hanno avanzato, nei diversi settori, una gamma molto ampia di proposte.

a sviluppare una politica e proposte solo dal lato della domanda e non anche dal lato dell'offerta. Non è così. E vi faccio rapidamente qualche esempio. esempio. Volete fare una politica anche dal lato dell'offerta e non solo dal lato della domanda? La norma che proponiamo - noi e voi, con i vostri emendamenti - sul trattamento fiscale degli affitti agisce contemporaneamente degli affitti agisce contemporaneamente dal lato della domanda, perché aumenta il reddito disponibile delle famiglie, e dal lato dell'offerta, perché, incrementando il mercato degli affitti, aumenta la mobilità del fattore lavoro sul territorio nazionale (scelta di tipo

questa è una norma di cui discutiamo da anni che, è vero, il primo anno ha un effetto pesante sulla finanza pubblica, effetto che però si riduce drasticamente nel secondo e nel terzo quando, secondo i calcoli di tutti,

nel senso che è tecnicamente provato che costa nei primi anni, ma che addirittura strategicamente produce un aumento del gettito a causa dell'emersione di quel gigantesco nero che nel settore degli affitti caratterizza il nostro sistema economico,

287.000 cantieri in Italia per piccoli interventi in abitazioni per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico. Le famiglie italiane stanno massicciamente investendo su questo versante. Abbiamo un effetto dal lato della domanda? Certamente sì, perché anche qui abbiamo reddito che si rende disponibile per le famiglie. Abbiamo un effetto dal lato dell'offerta? Clamorosamente sì, perché l'attività edilizia, che è bloccata,

Terzo esempio: detassazione certa e permanente, signor Vice Ministro, della quota di salario da contrattazione di secondo livello. Ma veramente voi pensate di poter andare a raccontare agli italiani che non ci sono risorse per farla? Abbiamo di fronte in questo caso il classico intervento che realizza effetti sia dal lato della domanda, perché parliamo di detassare i salari, e quindi certamente aumentiamo il potere d'acquisto del reddito dei lavoratori

più elevata è la produttività, più alto è il salario. Di conseguenza, interveniamo per affrontare una tabe dell'economia italiana degli ultimi 15 anni che è la costante caduta della produttività totale dei fattori e purtroppo, negli ultimi anni, anche della caduta della produttività del lavoro. Quarto ed ultimo esempio: detassazione dei redditi da lavoro femminile. È da considerarsi una politica dal lato della domanda? Certamente sì: sono redditi per lavoratrici che vanno nelle famiglie e quindi sostengono la domanda effettiva sotto il profilo dei consumi e sotto il profilo degli investimenti delle famiglie. Ma abbiamo anche qui un formidabile strumento di politica dal lato dell'offerta. Infatti, signor Vice Ministro, qual è la risorsa fondamentale in questo Paese per pensare di crescere a livelli significativi nei prossimi anni?

Per realizzare una crescita di questo tipo, qual è il fattore fondamentale produttivo inutilizzato esistente in Italia? La risposta è precisa: la straordinaria energia, capacità e disponibilità di lavoro di milioni di donne italiane, in particolare nel Mezzogiorno. Questa è la fondamentale risorsa per lo sviluppo del Paese nei prossimi decenni. Se detassiamo - con una misura che può partire piano e crescere nel tempo in modo significativo - il salario e i redditi delle donne

abbiamo un migliore utilizzo dei fattori produttivi, il che accresce - adesso ho poco tempo e lo devo dire con questo linguaggio incomprensibile - il prodotto potenziale del Paese. Se questi quattro esempi non sono inventati da un pazzo, ma sono esempi concreti di scelte politiche non particolarmente costose, che agiscono contemporaneamente dal lato della domanda e dell'offerta, allora: «*hic Rhodus hic salta*». La maggioranza si è confrontata, ha avuto ancora qualche giorno di tempo rispetto al dibattito in Commissione per arrivare a delle conclusioni. Non ci proponga degli ordini del giorno, per favore: ci proponga delle scelte!

vorrei innanzitutto ringraziare i relatori di maggioranza, Latronico e Saia, e quelli di minoranza, Morando e Mercatali per il lavoro svolto, e tutti i numerosi intervenuti a questo dibattito, che è stato molto ricco: credo dimostri come il Parlamento sia la sede opportuna per sviscerare seri problemi quando ve ne è l'occasione. L'occasione è anche quella per dire addio senza troppi rimpianti alla legge finanziaria, che ha accompagnato con una sorta di rito apotropaico i 30 anni scorsi della vita del nostro Parlamento, nel bene e nel male, ingigantendone le emozioni e liofilizzandone le responsabilità. È una morte annunciata, che non lascia rimpianti. Aspettiamo la prossima legge di stabilità, che credo potrà portare anche più razionalità al momento delle decisioni pubbliche in tema economico. Solo qualche considerazione di carattere generale, signora Presidente, tenendo conto che a quesiti specifici avanzati nel corso del dibattito mi riservo di rispondere quando si tratteranno gli emendamenti, principalmente riferiti alla legge finanziaria. Innanzitutto, una considerazione emersa dalla generalità dell'Assemblea, sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, ossia che il Governo ha avuto nella gestione della crisi economica una condotta corretta che ha portato a risultati positivi. Credo che debba essere valutato molto positivamente dal Governo il fatto che il Parlamento italiano gli dia questa sorta di viatico, tenendo conto che la crisi non è ancora del tutto terminata.

il sistema italiano ne esce stabilizzato, anche con le difficoltà che sono di fronte a tutti, principalmente nel settore dell'occupazione. Adesso, tuttavia, molte parti del Parlamento lamentano che il Governo si troverebbe davanti ad una sorta di immobilismo. Mi domando: è effettivamente immobilismo o si tratta di una travisazione dei fatti? In realtà, il Governo non è affatto immobile; basti vedere, per esempio, le iniziative assunte e le risorse stanziate: 18 miliardi nell'assestamento per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione; 8 miliardi aggiuntivi sulla cassa integrazione (che forse non vedrà strumenti giuridici perfezionati, però vede le erogazioni: quindi le situazioni dei singoli che sono in difficoltà alla fine vengono risolte); la massa d'urto che viene attuata con la Cassa depositi e prestiti e la SACE, che serve a dare garanzie alle imprese per andare in soccorso laddove il credito bancario è insufficiente, al fine di creare un sistema che garantisca alle nostre imprese, soprattutto quelle piccole e medio piccole, di andare avanti. molti effetti di grandi riforme che sono state attuate (forse un po' trascurate, come ad esempio quella del federalismo) non sono ancora visibili, ma arriveranno nel futuro e consentiranno di superare molte difficoltà. È un periodo di difficoltà in cui ci troviamo tutti.

un sorpasso in discesa, ma che sta a significare che le difficoltà sono comuni e il nostro Paese, che ha tradizionalmente maggiori difficoltà, riesce a resistere forse meglio di qualche altro Paese.

Mi domando se ciò nella realtà dei fatti del passato sia vero: l'esperienza, ahimè, dimostra che anche quando con le migliori intenzioni si è andati a diminuzioni della pressione fiscale riducendo la spesa, in realtà questa non si è mai ridotta veramente. Sono state adottate soluzioni, diciamo così, non sempre rigorose e, ahimè, la spesa pubblica è cresciuta negli anni. Quindi, anche ogni riduzione di imposte credo debba essere valutata secondo le categorie della realtà, considerando che, in effetti, malgrado le migliori intenzioni, spesso la diminuzione della pressione fiscale ha portato a corrispondenti aumenti di spesa. Per tale ragione in questo settore bisogna essere molto cauti. La tentazione in questo periodo di crisi o di post‑crisi è molto seria. Infatti, come dopo le due guerre mondiali gli Stati si sono trovati in possesso di maggiori risorse derivanti dall'aumento delle tasse per far fronte agli oneri di guerra e non le hanno restituite ai contribuenti, continuando ad utilizzarle per la spesa pubblica al fine di cercare un consenso che non sempre è arrivato, così la tentazione in questa fase di crisi, dove gli Stati hanno utilizzato e pubblicizzato molto più di prima l'economia, potrebbe essere quella di mantenere un rischio molto più grave della soluzione del problema. quindi porsi, in primo luogo, la domanda: come vogliamo che questo Paese si trovi dopo la crisi? Vogliamo un Paese in cui il *mix* tra l'economia pubblica e l'economia privata assomigli più a quello di un'economia di comando o vogliamo restare un Paese caratterizzato da libertà di mercato? Credo sia una domanda fondamentale

la perdita di capacità competitiva nel nostro Paese nello stesso periodo, forse possiamo dedurne un'equazione in base alla quale più spesa pubblica crea in realtà maggiori difficoltà allo sviluppo e non viceversa. Credo quindi che, non essendo dimostrato dal *New Deal* in avanti

sia valido esattamente il contrario. Ricordando un grande Presidente degli Stati Uniti, forse la spesa pubblica non è la soluzione del problema: la spesa pubblica è la causa di molti problemi. Ritengo pertanto sia indispensabile cercare di ridurre la spesa, ma per questo - appunto - non si devono trovare delle scorciatoie

una possibile uscita dalla crisi ma che non allontana tutte le nubi all'orizzonte, richiede una disciplina fiscale tanto più rigorosa quanto più difficile è la di perseguire una coesione sociale la più forte possibile, tanto più in un momento di difficoltà, per andare incontro alle persone che si trovano in maggiori avversità; richiede un sistema di sicurezza sociale

è proprio di oggi l'appello del presidente della Banca centrale europea Jean Claude Trichet, il quale sostiene che in questo momento di difficoltà, in cui è necessario consolidare i conti pubblici, i tagli delle tasse dovrebbero essere considerati - cito testualmente - «solo nel medio termine, quando i Paesi avranno di nuovo a disposizione sufficienti spazi di manovra a livello di bilancio».

assumendo un atteggiamento molto cauto in questo particolare settore. Certo, ciò non significa che se esistono storture - se, ad esempio, vengono tassate delle perdite - queste non possano essere corrette o che, se che, se nell'ambito delle disponibilità si può rivedere la tassazione, soprattutto riguardo ai soggetti più deboli - per esempio, alle piccole imprese -, alcune soluzioni non possano essere rinvenute. Intendo riferirmi tuttavia allo spazio di disponibilità per attuare una diminuzione della pressione fiscale, che se non fosse elevata non porterebbe effetti macroeconomici. Tutti i Governi - di questa e di quella parte - negli ultimi dieci anni si sono sforzati di operare delle riduzioni della pressione fiscale, ma tutti lo hanno fatto sostanzialmente al margine, e gli effetti economici sono stati sostanzialmente nulli. Pertanto, o la riduzione è molto cospicua o gli effetti non esistono. Tuttavia, perché una riduzione possa essere molto cospicua occorre trovare coperture molto serie che - non ci possiamo illudere - non possono che essere una riduzione della spesa pubblica nei grandi comparti sociali. È questa una soluzione possibile nell'attuale momento storico? Francamente avrei qualche dubbio. In conclusione, ringraziando ancora il Senato per l'appoggio che credo darà al Governo nell'opera volta ad assicurare una

ai sensi del comma 5 dell'articolo 129 del Regolamento, potranno intervenire su ciascun articolo unicamente i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli e quindi il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il rispettivo parere. Preciso che con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvati anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati nello stampato. Ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento, la votazione finale del disegno di legge di bilancio sarà effettuata solo dopo la votazione finale del disegno di legge finanziaria. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5aCommissione permanente sugli emendamenti presentati al provvedimento in esame. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

delle risorse per la giustizia. Il dato più clamoroso è rappresentato da due cifre: il fabbisogno stimato per il 2010 è di 8.380 milioni di euro,

di coprire le spese stimate per il prossimo anno senza avere in cassa circa un miliardo di euro.

l'estensione del gratuito patrocinio per le vittime di violenza sessuale, l'istituzione della banca dati del DNA, l'estensione dei casi di applicazione della misura cautelare in carcere e l'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel nostro Paese. Insomma, dalla lettura dei dati, considerato il bisogno di giustizia e di sicurezza che viene dal Paese il fatto che abbiamo assegnato alla giustizia un compito da volano

in aumento: quello relativo agli stipendi e agli assegni fissi di Ministro e Sottosegretari.

riguarda assegni e indennità di Ministro e Sottosegretari. Il Paese ha bisogno anche di risposte. Si dice che, purtroppo, questo è un settore che, come gli altri, subisce dei tagli, anche se il Paese ha bisogno di giustizia, di informatizzazione, di carceri, di sicurezza. Ma poi non si possono aumentare stipendi e indennità per Ministro e Sottosegretari. È un segnale negativo, impossibile da spiegare al Paese.

obbligatorie e fisse, quindi oneri inderogabili. I tagli ovviamente operano

le camere penali a proposito di ciò che in quest'anno e mezzo è stato fatto in materia di giustizia: «Molte «Molte delle novità, al di là del clamore mediatico artatamente alimentato sulla loro portata, costituiscono patrimonio già acquisito del cosiddetto diritto vivente; altre, invece, si candidano al ruolo di inutili, se non controproducenti orpelli che promettono solo di incidere negativamente sull'efficienza della macchina processuale». Questo è il dato sconfortante della nostra produzione legislativa cui si accompagnano i tagli, vigorosi, al sistema giustizia, che avrebbe invece bisogno di risorse, nell'interesse dei cittadini.

Si tratta di appostazioni diverse di somme non particolarmente rilevanti, ma qualitativamente significative.

al programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» e, ancora, un'analoga somma per il potenziamento delle attività relative al programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario». Non ho bisogno di argomentare l'importanza di potenziare lo sforzo in queste due direzioni. Abbiamo avuto modo di denunciare spesso la necessità di alzare la soglia di contrasto nella repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali.

efficacemente in questa direzione. Allo stesso modo la tematica della regolamentazione e della vigilanza sul settore finanziario, per le vicende che abbiamo conosciuto, richiede la massima sollecitudine e strumentazioni appropriate.

colleghi interverranno successivamente illustrando altri emendamenti in materia di ordine pubblico e di funzionamento del settore difesa. Mi limito semplicemente a richiamare l'attenzione sul fatto che anche la Guardia di finanza elemento di aiuto, di supporto, un contributo determinante nel campo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non ho bisogno di richiamare le esternazioni di ieri del ministro Maroni per dire quanto sia

a queste specifiche appostazioni di bilancio. Spero che quel parere, che non abbiamo condiviso per valutazioni di carattere complessivo, ma che su questo aspetto rifletteva esattamente le sollecitazioni e le proposte venute dall'opposizione,

potenziare l'apporto del Corpo al raggiungimento degli obiettivi di lotta all'evasione fiscale e contrasto dei reati finanziari e del riciclaggio e ritiene opportuno esaminare la possibilità di concentrare maggiormente le risorse definite nella tabella sui capitoli di spesa maggiormente correlati con la specifica attività di istituto, consentendo una maggiore premialità del merito e della produttività». È esattamente ciò che pensiamo, e che abbiamo tradotto in un emendamento che mi auguro possa trovare

e 2.Tab.2.43, unitamente ad altri successivi inerenti alle risorse per il comparto difesa e sicurezza. Gli emendamenti si prefiggono lo scopo di garantire finanziamenti adeguati al settore dell'esercizio e del funzionamento, che costituiscono la base operativa delle nostre Forze armate e delle forze di Polizia. Si riferiscono, infatti, alle esigenze di manutenzione di tutti i mezzi e dei sistemi d'arma, di adeguamento delle infrastrutture, di approvvigionamento delle scorte, di tutti i materiali e dei ricambi. Si riferiscono, ancora, al funzionamento dei centri tecnici e dei poli logistici, nonché degli arsenali della marina, ma soprattutto si riferiscono alle attività relative all'addestramento e alla formazione del personale militare e di polizia, che risulterebbero fortemente penalizzate dalle assegnazioni finora previste. Tutti i colleghi senatori sono pienamente coscienti del forte impegno delle Forze armate e delle forze di Polizia. Sanno che quelle forze sono chiamate continuamente ad intervenire, all'estero per il mantenimento della pace, in Italia per il controllo del territorio o nel contrasto alla criminalità o in soccorso delle popolazioni colpite da pubbliche calamità, o ancora in tante altre circostanze. E sanno che quelle forze hanno sempre dato una risposta pienamente soddisfacente, di cui tutti ci siamo sentiti e ci sentiamo orgogliosi. Sono convinto, pertanto, che sia intendimento di tutti noi mantenere alta l'efficienza operativa e logistica dei comparti difesa e sicurezza. D'altro canto, non sono solo io a chiederlo, né è solo il Partito Democratico: è stata la Commissione difesa del Senato che più volte ha ricordato l'esigenza di garantire risorse adeguate per l'efficienza del comparto. Sono stati i Capi di stato maggiore della Difesa e delle singole Forze armate a sottolineare il pericolo derivante da una insufficiente disponibilità di risorse. Sono stati gli operatori della sicurezza, con l'imponente manifestazione di qualche giorno fa, a ricordarci il loro disagio professionale. Sono stati infine gli stessi Ministri della difesa e dell'interno a ribadire frequentemente, e in circostanze diverse, che i comparti devono poter contare su finanziamenti sicuri soddisfacenti. Allora, signori senatori, operiamo per venire incontro alle legittime richieste del comparto. Certamente non saremo in grado di avvicinare, per esempio, la percentuale del PIL dedicata alla nostra difesa, che attualmente è allo 0,90 ai valori medi dei Paesi europei con i quali ci confrontiamo, che sono all'1,42 per cento, ma quanto meno evitiamo di rendere più difficile alle nostre Forze armate armate e alle forze di Polizia l'assolvimento di quei delicati compiti ai quali cui esse sono totalmente e generosamente dedicate. Gli emendamenti presentati dal Partito Democratico si prefiggono solo questo scopo. Per questo mi auguro fortemente che la maggioranza e il Governo vogliamo esprimere nei loro riguardi un parere favorevole: un parere favorevole che sarebbe il concreto riconoscimento della loro funzione e non un vuoto *spot*, come molto spesso accade.

la competitività e lo sviluppo delle imprese, con particolare riguardo agli interventi per il Mezzogiorno. I nostri emendamenti, in particolare, si soffermano sulla necessità

e che non va nella direzione - come pur sarebbe auspicabile e condivisibile da parte nostra - di tagliare spese improduttive. Al contrario, si taglia ad esempio per 16 milioni di euro il Fondo per gli interventi agevolati alle imprese; per ben 92 milioni di euro il Fondo per la competitività e lo sviluppo delle imprese; per 13 milioni di euro il Fondo rotativo per le imprese; per 8 milioni di euro il Fondo per la concessione del credito d' imposta per l'occupazione nelle aree sottoutilizzate;

e che invece viene sostanzialmente prosciugato nelle sue risorse. Insomma, attorno a questa missione e a questo capitolo di spesa, siamo in presenza di una sostanziale riduzione di risorse e di un annullamento di questi interventi assolutamente non improduttivi e quindi fondamentali per le politiche di sostegno al sistema delle imprese, in particolare nelle aree sottoutilizzate.

con l'emendamento 2.Tab.2.45 sulla missione «Sviluppo e riequilibro territoriale». Con quella misura, infatti, anche qui abbastanza inopinatamente, si tagliano e si annullano del tutto le risorse

Zanda. Essi riguardano tutti lo stesso tema e cioè la necessità, secondo noi urgente e vitale per il nostro Paese, di ripristinare le risorse decurtate con questo bilancio al Ministero dell'ambiente. Lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2010 reca spese per circa 740 milioni di euro, con una riduzione del 42,6 per cento rispetto alle previsioni assestate del 2009. In particolare, gli stanziamenti attribuiti alla missione principale del Ministero dell'ambiente, la missione 18 («Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente») si dimezzano, passando da 1.112 a 595 milioni. appare di assoluta gravità - per ragioni evidenti, credo, a tutti i colleghi - la fortissima riduzione delle previsioni di spesa in un campo, quello della conservazione dell'assetto idrogeologico, che riguarda uno degli aspetti di più acuto degrado dei nostri sistemi ambientali. Esso

prima con il terremoto dell'Aquila, poi con la tragedia di Messina, è stata confermata la condizione di insicurezza abitativa in cui vivono centinaia di migliaia di italiani, collegata al rischio sismico e idrogeologico, ma largamente alimentata da un uso spesso distorto del territorio. Ebbene, al termine di un anno come questo, nel bilancio di previsione per il 2010 gli stanziamenti per la difesa del suolo toccano il loro minimo: dai 510 milioni dell'ultima finanziaria del Governo Prodi si è passati ai 270 milioni del 2009 e ai 120 milioni previsti per l'anno prossimo. in particolare, viene del tutto azzerato lo stanziamento relativo ai piani strategici per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento del territorio, da attuare d'intesa Ritengo che questo sia uno dei capitoli più infelici del bilancio che ci accingiamo a votare e di più palese contraddizione con le necessità del nostro Paese. Fino ad ora, il Ministro dell'ambiente ha strillato un po', ha detto che queste risorse non bastano quasi nemmeno all'ordinario funzionamento del suo Ministero, ma - come spesso le è capitato da quando ha assunto questa responsabilità - i suoi strilli si sono fermati nell'anticamera del Consiglio dei ministri, almeno per quello che è dato di capire. Con i nostri emendamenti, noi cerchiamo di porre un parziale rimedio a questa decurtazione di fondi. L'Italia di tutto ha bisogno, credo, tranne che di vedere ridotte così drasticamente

Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, illustrerò alcuni emendamenti che riguardano il tema della sicurezza e della mobilità

il numero degli incidenti in cui restano coinvolti ciclomotori e motoveicoli, che si verificano annualmente sulle strade urbane ed extraurbane, malgrado i tentativi di ridurne la portata, non accenna a diminuire in misura significativa. legislativo n. 285 del 1992, prevede che le norme e i provvedimenti attuativi si ispirino al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico e di migliorare il livello della qualità, cioè una serie di cose che potrebbero accadere solo se ci sono le necessarie risorse.

voglio dire a tutti che è indispensabile un incremento degli stanziamenti. Nella fattispecie, proponiamo un aumento di 35 milioni di euro, sia per competenza che per cassa, proprio per intervenire su questo versante. sul tema della mobilità pubblica locale. È un sistema che, nella sua efficienza e nella sua necessità, dovrebbe dare risposte concrete, ma anche in questo caso c'è una mancanza di sensibilità da parte del Governo. Nonostante la mobilità locale mostri una realtà davvero drammatica, anche in tale comparto troviamo una riduzione degli stanziamenti, che chiediamo vengano incrementati per 20 milioni di euro, destinati allo sviluppo della mobilità locale e del programma del Ministero delle infrastrutture.

mostrano ancora una volta che la povertà e la disuguaglianza continuano ad essere un problema rilevante nel nostro Paese. Tra i Paesi dell'Europa «a 15», la situazione italiana è ancora tra le peggiori, insieme a quella

mentre gli individui poveri sono 7.537.000. Oltre alla grave situazione delle famiglie i cui componenti hanno perso il lavoro, sempre più difficoltà incontrano quelle famiglie che, pur avendo un reddito, non riescono a far fronte a tutte le spese mensili minime necessarie per la sussistenza e per l'abitazione. Per Per compensare questa variazione negativa, chiediamo di incrementare di 5 milioni di euro il capitolo che riguarda la spesa inerente alla casa e all'assetto urbanistico, proprio per rafforzare le politiche urbane e territoriali di questo Paese.

come ampiamente emerso dal dibattito, il disegno di legge recante la manovra finanziaria per l'anno 2010 non sembra francamente rispondere alle esigenze primarie del nostro Paese e lascia disattesi tutti i grandi progetti di sviluppo infrastrutturale. Dalla manovra di bilancio emerge una realtà ben diversa da quella che il Governo, sin dall'inizio della legislatura, ha più volte manifestato con l'intenzione di voler contribuire in maniera significativa allo sviluppo del sistema infrastrutturale del Paese. I tagli di spesa colpiscono vari settori e gli emendamenti che abbiamo presentato hanno lo scopo di dare almeno un timido segnale di riequilibrio. In particolare, gli stanziamenti relativi al diritto alla mobilità, alle infrastrutture pubbliche e logistiche e alla casa e assetto urbanistico, che insistono in tabella 2, sono stati drasticamente ridotti. Per quanto attiene al diritto alla mobilità, il Governo opera una riduzione di 3.352 milioni di euro, rispetto agli 8.086 milioni di euro delle previsioni assestate 2009, le principali riduzioni riguardano le somme da assegnare alle Regioni per opere di adeguamento stradale, che passano da circa 5,5 miliardi a poco più di 3 miliardi. I contributi alle Ferrovie dello Stato

del programma «Sviluppo della mobilità locale» è stato effettuato un pesante taglio pari a 380 milioni di euro per l'anno 2010, di cui 124 milioni a riduzione delle risorse disponibili per i rinnovi per i rinnovi contrattuali del trasporto pubblico locale, 100 milioni di euro per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi del trasporto pubblico, 50 milioni di euro per elevare il loro livello di sicurezza, altri 50 milioni per la realizzazione del trasporto rapido di massa a guida vincolata e tranvie, e 48 milioni di euro per favorire la realizzazione di sistemi ferroviari passanti. Con gli emendamenti presentati ne riproponiamo l'allocazione di almeno un quarto, consapevoli degli effetti che si produrranno in termini di conflittualità e disagio a livello locale. Con riguardo al programma delle politiche abitative, viene previsto un taglio di 207 milioni di euro rispetto alle previsione assestate, di cui oltre 37 milioni di euro per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Il taglio del contributo in conto affitto è purtroppo una costante: noi contribuiamo a metterlo e il Governo di centrodestra sostanzialmente lo toglie. Forse varrebbe la pena mettersi d'accordo, magari anche conoscendo meglio il problema. Viene soppresso il capitolo relativo all'edilizia sperimentale, che recava 104 milioni di euro. I contributi ai Comuni passano da 204 a 164 milioni di euro. I tagli hanno colpito anche il piano nazionale di edilizia abitativa, con la riduzione di oltre 20 milioni di euro. Com'è evidente, da quando il piano casa, grazie al contributo delle Regioni titolari delle competenze in materia, è divenuto una cosa un po' più seria, l'attenzione al riguardo da parte del Governo è durata davvero lo spazio di un sorriso. Mi riprometto di intervenire in dichiarazione di voto per quanto riguarda i pesanti tagli fatti al sistema infrastrutturale del nostro Paese, segnatamente sui porti e sugli aeroporti, che sono i nostri principali *gate* naturali per passeggeri e merci.

proposte emendative sono finalizzate a reintegrare gli stanziamenti tagliati alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese» e in particolare al programma «Regolamentazione e incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale». Si tratta di un taglio lineare di 84 milioni di euro circa, che colpisce il contributo statale a progetti in favore di distretti produttivi adottati dalle Regioni e di carattere nazionale; colpisce il fondo per investimenti agevolati alle imprese e azzera il fondo per il finanziamento per il salvataggio delle imprese in difficoltà. Mi sembra che il Governo e la sua maggioranza in materia di politica economica, e in particolare di politica industriale, in questo caso siano incoerenti, perché se da una parte fanno dichiarazioni ufficiali circa l'importanza delle piccole e medie imprese per la ripresa dell'economica e dell'occupazione nel nostro Paese, dall'altra non solo non intervengono con misure efficaci e anticicliche, ma allo stesso tempo apportano tagli rispetto alla previsione dell'anno passato su voci di bilancio molto importanti per le stesse PMI. In particolare, tenere sotto controllo i conti pubblici non significa fare tagli generici che, oltre ad essere inefficaci, sono anche dannosi. Penso al taglio operato sui contributi per i distretti produttivi in questo caso, che sono in crisi perché hanno perso fatturato e quote di mercato soprattutto verso l'estero, e in particolar modo al fatto che la legge n. 99 del 2009 in materia di sviluppo economico, approvata con il contributo di tutte le forze politiche, ha previsto alcune norme che volevano dare una risposta al mondo produttivo, che chiede ormai da tempo condizioni di contesto che favoriscano processi di innovazione per uscire dalla crisi. Per questo abbiamo previsto accordi di programma, per gli interventi di reindustrializzazione delle aree e dei distretti in crisi; l'agevolazione delle relazioni di filiera e di rete attraverso una norma che prevede il riconoscimento giuridico delle reti di impresa come modello di aggregazione innovativo, anche per convogliare poi i finanziamenti pubblici. Tuttavia, se non vengono stanziate risorse per attivare queste misure, o ancora di più se si prevedono tagli importanti a queste missioni dirette a finanziare

questo prodotto, che noi riteniamo la chiave di volta del nostro sviluppo economico. Mi chiedo quando si potrà con efficienza dare seguito a queste misure, visto che le risorse sono tagliate in modo consistente.

Signora Presidente, cercherò di essere breve per essere compatibile con gli orari degli aerei, visto che è cosa prioritaria.

all'estero. Sui sette capitoli per le comunità italiane all'estero nella finanziaria 2008 erano previsti e messi a disposizione 58 milioni di euro.

non puntano e non mirano a tornare ai livelli del 2008, che erano comunque già molto stretti, ma a mantenere semplicemente per il 2010 la stessa disponibilità che si è avuta per il 2009.

si può insegnare l'italiano ai discendenti dei nostri emigrati. Con 6 milioni si chiede poi di far fronte ai destini non sempre di successo di emigrati nati in Italia che in America Latina vivono in stato di indigenza. Chiedo, cari colleghi - soprattutto a quelli della maggioranza, che seguono con interesse e con impegno

che si vogliono piantare, perché l'obiettivo è mantenere il livello minimo che abbiamo avuto per il 2009. Credo che il relatore ed il Vice Ministro possano dare un parere positivo su queste due minime richieste. Non c'è alcuna volontà di tornare a finanziamenti non compatibili con la politica di questa maggioranza. Semplicemente si chiede di mantenere i livelli del 2009. Dare una risposta adesso, Vice Ministro, vuol dire non tornare con una richiesta in assestamento di bilancio e, soprattutto, garantire un utilizzo estremamente più razionale di queste poche risorse da parte del Governo e dell'amministrazione. Mi auguro che su questi modestissimi emendamenti si possa dare un segnale agli italiani all'estero che in questo momento fanno una gran fatica a mantenere alta la nostra immagine nel mondo. Vorrei concludere su un fatto di questi ultimi giorni. L'Agenzia delle entrate ha spedito, soprattutto in Svizzera, ai frontalieri, decine di migliaia di lettere

una tale contraddizione che voglio semplicemente definirlo un errore, una distrazione dell'Agenzia delle entrate. Questa mattina con i colleghi

chiedere a dei lavoratori emigrati di dover scudare la loro pensione o il loro stipendio. Si tratta, mi auguro, di un errore. Ripeto, ci aspettiamo da parte del Governo e del relatore una risposta la prossima settimana in finanziaria.

*(PD)*. Presidente, vorrei mettere in luce con questi emendamenti che un servizio efficiente della giustizia può essere fornito soltanto se si procede all'attribuzione di maggiori risorse ad un settore così cruciale, cui è destinato solo l'1,6 per cento delle risorse complessive del bilancio dello Stato; risorse che sono state già ridotte nel 2008, decurtate nella misura del 40 per cento Interveniamo con questi emendamenti su settori delicatissimi, che sono la giustizia minorile, la giustizia penitenziaria, le spese correnti dell'amministrazione. È evidente che il complessivo aumento del numero dei reati ed oltretutto l'ipotesi di cattura obbligatoria, che aumentano anche la fase della custodia cautelare e delle detenzioni definitive, creano un problema molto serio, perché la mancanza di risorse non consente di rispondere adeguatamente ad un servizio giustizia che non soltanto deve essere efficiente per la giustizia stessa ma anche per la sicurezza.

la mobilità, la sicurezza, i distretti produttivi: tutti programmi di spesa che, presi singolarmente, ovviamente meritano considerazione e di cui credo che il Governo non potrà non tener conto. i singoli stanziamenti vanno inquadrati nella fisionomia e nell'assetto del bilancio e, dovendo mantenere i saldi (di cui abbiamo parlato) il mio parere non può che essere

esige che vi sia un lavorio all'interno delle Commissioni di merito per vedere se la dislocazione della spesa all'interno di un programma per missioni effettivamente corrisponda a quegli indicatori di *performance* che potrebbero consentire magari una riallocazione. Vi è quindi un problema di responsabilità che il Parlamento ha dinanzi a sé, le singole Commissioni di merito possono lavorare meglio sugli stanziamenti disponibili, per portare avanti quel percorso di revisione che ci metta in condizione, intanto, di utilizzare in maniera efficace le risorse di cui disponiamo, e anche - perché no? - di utilizzare un lavoro sistematico, non solo nella sessione del bilancio, per verificare nelle singole Commissioni di merito l'idonea ed efficace distribuzione della spesa pubblica.

non dico obbligatorie dal punto di vista formale, ma sostanzialmente necessarie. Quindi, ciò significherebbe un aumento della spesa anche per far fronte a questioni rilevanti. far presente due corollari. In primo luogo, a volte nell'illustrazione degli emendamenti si è detto che essi servono a ripristinare il livello di spesa dell'esercizio precedente, il che potrebbe essere ragionevole, se non fosse che, rispetto all'esercizio precedente, è cambiato il mondo. Pertanto, se l'anno scorso avevo, ad esempio, uno stipendio molto elevato e questo anno ce l'ho più basso, devo adeguare il mio livello di spesa rispetto alle mie reali possibilità. il bel tempo perduto è bello, ma forse, per certi aspetti, è anche perduto. In secondo luogo, con la riforma del bilancio il Parlamento si potrà appropriare molto di più di prima di un potere di controllo reale sulla gestione della spesa,

alle amministrazioni di spesa in primo luogo, ma soprattutto al Parlamento, di valutare la congruità della spesa e quindi di fare uno lavoro di fino, una sorta di *fine tuning*, all'interno del bilancio, cosa che potrà essere svolta grazie. Sulla questione dei frontalieri, sollecitata con molto vigore, è ovvio che le entrate dei frontalieri che derivano dal lavoro non rientrano nella categoria dei

**Il Senato non approva.**

che abbiamo presentato contestualmente al sistema giustizia e al comparto sicurezza (perché riteniamo che siano due facce della stessa medaglia). In questa sede, in questo momento, dobbiamo parlare soltanto di tagli, e a questo ci limitiamo,

disegni di legge che voi non avete mai esaminato, che noi abbiamo sottoposto alla valutazione del Ministro della giustizia nel dicembre 2008 - quindi circa un anno fa

significativo la missione Giustizia e che sono suscettibili di determinare un ulteriore forte decremento dello standard qualitativo dell'amministrazione della giustizia, il rischio di arrivare addirittura ad una sua paralisi, ove si consideri che a questa missione sono ricondotti quattro programmi cruciali per la funzionalità della macchina giustizia e, quindi, anche per la sicurezza e la tutela dei diritti dei cittadini. come quelli dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia civile e penale, della giustizia minorile e dell'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile; «Giustizia» fortemente penalizzato appare il programma «giustizia civile e penale», che subisce i tagli di spesa più gravi (oltre i 429 milioni di euro); viene così colpito il funzionamento ordinario dell'amministrazione della giustizia. In particolare riguarda il settore penitenziario, ricordo che la riduzione delle risorse previste per il Ministero della giustizia non solo non consentirà di affrontare l'emergenza che caratterizza la situazione attuale del sistema penitenziario ma aggraverà ulteriormente la condizione di sovraffollamento, disfunzionalità e disagio che si riscontra in molte delle carceri italiane che ospitano un numero di persone di molto eccedente rispetto alla capienza regolamentare, di grave rischio per l'incolumità e la sicurezza dei detenuti e degli stessi agenti di polizia penitenziaria. Infine, le forti riduzioni di spesa previste dal Ministero della giustizia ostacoleranno in misura significativa la piena attuazione delle politiche per la sicurezza e il contrasto alla criminalità, impedendo il celere ed effettivo accertamento dei reati e l'identificazione dei colpevoli, nonché la prevenzione dei delitti, in palese contraddizione con quanto asserito dagli esponenti del Governo e della maggioranza non solo in sede parlamentare o in contesti istituzionali ma anche nell'ambito di dichiarazioni rese pubblicamente ai mass media.

per sottolineare una questione per la verità amplificata dalle dichiarazioni rese ieri dal Ministro dell'interno in un incontro con i sindacati di Polizia. Se non ricordo male, ieri il Ministro dell'interno ha detto che se le opposizioni avessero presentato emendamenti funzionali all'incremento dei capitoli di bilancio relativi alla sicurezza, il suo partito, la Lega, avrebbe votato a favore.

di identificazione e di espulsione, che è stato bocciato. Onde evitare che vengano bocciati anche questi due ulteriori emendamenti (uno all'incremento di 150 milioni di euro per il contrasto alla criminalità interna ed internazionale, alla mafia, alla camorra, alla 'ndrangheta il potenziamento dei servizi di contrasto all'immigrazione clandestina, alla gestione delle banche dati ai fini della sicurezza e altre attività di misure di prevenzione generale; che prevede un ulteriore stanziamento di 150 milioni di euro per la pianificazione e la programmazione generale dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, per la pianificazione e il coordinamento delle attività finalizzate al potenziamento e all'ammodernamento delle strutture, alla ricerca scientifica e tecnologica, alle misure a tutela dei testimoni di giustizia e dei collaboratori di giustizia, per le vittime del dovere, per le attività investigative e le operazioni speciali) segnalo ai colleghi della Lega grazie.

che ci sono emendamenti che se votati potrebbero fare qualcosa di più e di diverso per le nostre forze dell'ordine e per il contrasto alla criminalità organizzata e comune: per la prima volta, qualcosa di concreto e non uno spot. Chiedo

le dotazioni del Fondo per le politiche sociali, tagliate per quasi 300 milioni e, infine, il Fondo per la non autosufficienza, interamente azzerato rispetto alla dotazione precedente di 400 milioni.

grazie.

Abbiamo fatto i conti anche noi: quella richiesta era giusta ed era non solo proporzionata, ma valeva soprattutto a controbilanciare i dati - che sono oggettivi e inequivocabili - secondo cui, con le ultime due manovre finanziarie, a partire dal 2008 e sino al 2010, vengono tagliati, soltanto sul Ministero dell'interno, 900 milioni di euro destinati alla sicurezza. Per il 2011 il taglio che si annuncia e che rimane inalterato è di oltre 492.000 milioni di euro.

Alle dichiarazioni del ministro Maroni sono seguite le dichiarazioni del ministro La Russa, perché quando parlo di tagli pari a 900 milioni di euro mi riferisco esclusivamente al Ministero dell'interno e non valuto quelli operati al Ministero della difesa e al Ministero della

il Governo e la maggioranza stanno ancora alla fase dell'analisi e, comunque, questa analisi non mi pare produttiva di misure che ci auguriamo intervengano; se non altro, perché il tema della sicurezza è stato uno dei tratti distintivi della campagna elettorale e del Governo Berlusconi,

al Senato e alla Camera sono stati caricati della dichiarata volontà e ferrea determinazione del Governo di intervenire a tutela della sicurezza dei cittadini. Il fatto è che si sono fatte molte chiacchiere e nessun fatto. fatto. Al contrario, se andiamo a guardare i conti, essi testimoniano indubitabilmente che il Governo ha ritenuto di tagliare una cifra ingente ‑ anzi direi ingentissima - sulla sicurezza, al punto che lo stesso Ministro dell'interno e il Ministro della difesa si trovano in una situazione di vera difficoltà, di fronte ad una sollevazione cui hanno dato voce anche tutti i sindacati di polizia e ad un disagio sempre più evidente della popolazione,

il ministro Maroni ha detto ieri, in un momento di risentimento e di verità politica che comprendiamo pienamente, che se ci fossero stati emendamenti dell'opposizione li avrebbe votati e accolti.

territori a fronteggiare anche le proteste del Paese e degli operatori della sicurezza - introducendo un principio di discussione su questo tema, che è caro a noi, nonostante l'irrisione che spesso ci è venuta dai vostri banchi, almeno quanto è caro alla maggioranza e al Governo, penso che faremo una buona cosa. Lo dico chiedendo il voto su questo emendamento, e lo ripeteremo per tutti quegli emendamenti della finanziaria che riguardano questo tema.

in fatti e invitiamo i colleghi della maggioranza a mostrare quantomeno un segno di disponibilità anche perché - lasciatemelo dire - lo facciamo per il vostro bene.

- le dichiarazioni del nostro Ministro per valorizzare il merito e la qualità e per fare in modo che le università possano addirittura essere concorrenziali tra di loro, perché siano i giovani a scegliere la migliore università e i migliori corsi. senza un diritto allo studio implementato, i ragazzi sceglieranno l'università più vicina a casa, a prescindere dalle motivazioni, dalle inclinazioni o dalle attitudini.

Con questa decisione del Governo viene archiviata la lotta al *digital divide* (ricordo che sono milioni gli italiani oggi esclusi da Internet) diventa impossibile la modernizzazione della pubblica amministrazione promossa dal ministro Brunetta e ci si priva, inoltre, di una misura importante di politica industriale di contrasto alla crisi economica. Con il nostro ordine del giorno vogliamo chiedere al Governo un ripensamento. Voglio ricordare che con il *budget* di 800 milioni previsto si possono mobilitare risorse di circa 1,4 miliardi di euro per lo sviluppo della banda larga. Ricordo che senza questo piano rinunciamo ad un incremento di PIL di oltre 2 miliardi di euro; rinunciamo ad assumere 4.000 ingegneri, 11.000 tecnici, 6.000 impiegati, 28.000 operai. Questi sono i dati del Governo sul progetto del vice ministro Romani. Soprattutto, rinunciamo alla modernizzazione del settore delle telecomunicazioni e quindi ad un vero incremento della produttività delle nostre imprese. In questo modo il Governo non investe sul futuro, in questo modo l'Italia rimane ultima della classe in Europa per gli accessi a Internet; in questo modo l'Italia uscirà più tardi e più debole e più debole dalla crisi economica attuale. Per queste ragioni chiediamo al Governo un ripensamento su tale piano, peraltro promosso dal Governo stesso, per scongelare questi fondi e dare all'Italia la possibilità di tornare ad essere tra i primi della classe in Europa e nel mondo sui temi dell'innovazione tecnologica. sono stati presentati diversi ordini del giorno. Illustrerò brevemente soltanto quello relativo al *made in Italy* che mi sembra il più significativo;

l'ordine del giorno che abbiamo presentato, il G3.108, va in questa direzione. Chiediamo al Governo che ripristini risorse che sono state sottratte,

La crisi economica internazionale ha prodotto effetti molto gravi sulle imprese del *made in Italy*. Solo 11 dei 104 distretti riconosciuti in Italia hanno registrato nel secondo trimestre del 2009 un aumento dei valori esportati; si chiude con un nuovo forte calo delle esportazioni (meno 26 per cento); per il settimo trimestre consecutivo le esportazioni non crescono o si contraggono e si prevede una situazione ancora più grave per i distretti del Mezzogiorno, dove il tema della competitività presenta ulteriori problemi irrisolti. Oggi più che mai è necessario che le nostre imprese siano sostenute nella fase di apertura dei nuovi mercati nei paesi emergenti perché, nonostante i rischi e la crisi, le aziende esportatrici del *made in Italy* possano combattere ad armi pari, in un mercato sempre più fondato sulla competizione. In una fase di recessione dell'economia mondiale e di crisi dei mercati finanziari è fondamentale il rifinanziamento degli strumenti di agevolazione del credito all'esportazione, mentre il Governo con la legge di bilancio taglia le già esigue risorse, con il pericolo di pesanti danni per le imprese italiane esportatrici di beni di investimento. Con questi ordini del giorno chiediamo il sostegno concreto ai distretti produttivi e alle esportazioni, indicando l'assoluta incongruenza dei tagli rispetto alla situazione delle piccole e medie imprese italiane. Sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il 2010 c'è un taglio di oltre 222 milioni di euro alla missione: "Competitività e sviluppo delle imprese". Il taglio colpisce in modo particolare i progetti in favore dei distretti produttivi, il Fondo per gli interventi agevolati alle imprese, senza contare l'azzeramento delle risorse per il salvataggio delle imprese in difficoltà,

Però credo non si possa continuare a lavorare così e che il rispetto nei confronti dei colleghi sia comunque dovuto.

qui ne va anche del diritto di ogni singolo collega di poter parlare in un'Aula silenziosa; è una questione di dignità del Parlamento. Altrimenti sospendo la seduta un quarto d'ora e poi riprendiamo. Lo so che non è bello, allora non costringetemi a gesti che non fanno parte della mia cultura. Sin quando l'Aula non sarà silenziosa, noi non riprenderemo a lavorare.

non credo che abbia cose super importanti perché si riduce di circa 22 milioni di euro lo stanziamento per l'anno 2010 relativo alla missione «Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo»; in tale ambito i tagli operano sull'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero e a ciò si aggiungono i tagli relativi alla promozione del *made in Italy* (17 milioni di euro in meno in termini di competenza). Gli ordini del giorno indicano quindi la necessità di una radicale correzione di rotta, chiedendo l'impegno del Governo nel ripristinare le risorse tagliate per il 2010 e predisporre per gli anni 2011 e 2012 adeguate misure per il sostegno della competitività delle imprese e per garantire il mantenimento almeno degli attuali livelli occupazionali.

Signor Presidente, colleghi, gli ordini del giorno vanno tutti nella direzione di dare impulso al Governo su materie importanti e significative che riguardano il *made in Italy*, l'internazionalizzazione e il *digital divide*, una serie di temi che credo rappresenteranno uno spunto ed un impulso per il Governo e per la sua azione di programmazione e anche di legislazione. Esprimo pertanto

Vorrei anche aggiungere che stiamo parlando di alcuni miliardi pagati dai lavoratori e dalle imprese che non sono tornati ai lavoratori e alle imprese sotto forma di prestazioni della cassa integrazione guadagni.

Si parla tanto, da parte del Governo, di accelerare i tempi della giustizia nei procedimenti sia civili che penali, di piena implementazione del processo telematico e di completa informatizzazione degli uffici, e poi, quando si chiede un impegno specifico, si dicono soltanto parole, senza

testualmente dichiarato che non ci sono le risorse al suo Ministero per fare un piano strutturale organico di contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e che

Le ragioni di fondo che hanno informato queste nostre iniziative risiedono nel fatto che il Governo, oltre ad aver scelto di trascurare vergognosamente l'ambito della sicurezza, ha assunto analoga decisione per quanto riguarda l'ambito della difesa, delle Forze armate, tant'è che noi sia nell'emendamento sia negli ordini del giorno chiediamo che venga disposto uno spostamento di risorse a favore dell'addestramento, della manutenzione dei mezzi e della sicurezza del personale. Abbiamo allargato il discorso alla dotazione degli organici, tenuto conto del fatto che circa 4.000 militari precari con certezza dovranno abbandonare il loro lavoro dopo sei-sette anni di attività, e abbiamo inoltre chiesto la realizzazione dei piani industriali.

ha ritenuto ‑ debbo supporre questo ‑ di non dover inserire nel disegno di legge finanziaria il capitolo di spesa relativo alle missioni internazionali.

fronte agli operatori agricoli che stanno manifestando in tutte le piazze italiane: siete voi che avete promesso il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale; siete voi che avete promesso il Fondo irriguo; siete voi che avete promesso il rifinanziamento delle agevolazioni; siete voi che avete promesso misure specifiche per questo settore. Solo una settimana fa la Francia ha concesso un miliardo di euro di finanziamenti per il settore agricolo. Ciò significa che in Europa adesso la nostra agricoltura è povera, ma sarà ancora più povera e meno competitiva nel futuro. Per

su una questione importante. Il senatore Gasparri, che ringrazio per questo, ha fatto circolare un'interrogazione relativa allo studente iraniano Mahmud Vahidnia, che spero tutti abbiamo sottoscritto. bisognerebbe chiedere al Governo se intende mantenere aperta la propria ambasciata a Teheran, come ha fatto durante le manifestazioni degli studenti, affinché, visto e considerato che - ahinoi - le manifestazioni represse con la violenza proseguono, si possa continuare a dare in qualche modo aiuto a chi manifesta senza l'uso della violenza a Teheran ed eventualmente concedere dei visti urgentemente per farli venire in Italia. **Per

Signor Presidente, volevo solo ricordare che domani si svolgerà la Conferenza nazionale sull'amianto e che noi abbiamo presentato, a tutela dei lavoratori ex esposti ad amianto, tutta una serie di interrogazioni, sollecitate più volte, cui il Governo non si è degnato di rispondere, neanche in Commissione. Quindi, per rispetto nei confronti degli ex lavoratori